L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

con il termine favismo, che ritengo ben noto ai presentatori, si indica un difetto congenito di un enzima, il glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), normalmente normalmente presente nei globuli rossi, essenziale per la vitalità funzionale degli eritrociti e, soprattutto, per i processi ossidoriduttivi che in essi si svolgono, legati alla loro capacità di assumere e veicolare ai tessuti l'ossigeno indispensabile alle funzioni vitali. Fino al 1° agosto 2007 non era consentito *sic et simpliciter* l'accesso nelle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ai soggetti carenti, in forma parziale o totale, di tale enzima. Successivamente, in considerazione di nuove risultanze e nuove tecnologie nel campo diagnostico e in quello della ricerca scientifica, si è ritenuto opportuno riconsiderare la compatibilità di alcune patologie che di per sé non possono essere aprioristicamente fattore di discriminazione - al fine della valutazione medico-legale dell'idoneità per l'espletamento del servizio militare. Come è noto, una commissione scientifica allo scopo istituita ha stabilito che i soggetti affetti da favismo nel senso sopra citato possono essere considerati abili a svolgere le attività connesse con lo *status* di militare secondo un principio di gradualità, ossia prevedendo opportune prescrizioni in relazione alla carenza di G6PD, per particolari attività. Sulla base di tali risultanze, considerata la necessità di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità, sono stati emanati due decreti dirigenziali (che hanno apportato modifiche agli analoghi strumenti normativi) e la discendente direttiva applicativa, i cui principi essenziali si sostanziano in due punti, il primo dei quali è l'idoneità al servizio militare incondizionato per gli di sesso maschile con attività G6PD maggiore o uguale al 30 per cento e per quelli di sesso femminile con attività G6PD maggiore o uguale al 70 con attribuzione di un coefficiente di idoneità pari a 2, che esprime una condizione di assenza di patologia, ovvero una presenza di situazione sanitaria compatibile con l'espletamento del servizio militare incondizionato. Tali soggetti, idonei al servizio militare incondizionato, possono essere arruolati in tutte le categorie di personale (ufficiali, sottufficiali, volontari di truppa in servizio permanente e volontari di truppa in ferma prefissata) continuando ad esistere alcune specifiche precauzioni in caso d'impiego in zone malariche. Il secondo punto è l'idoneità al servizio militare per gli individui di sesso maschile con attività G6PD inferiore al 30 per cento e per quelli di sesso femminile con attività G6PD inferiore al 70 con l'attribuzione di coefficienti pari a 3 e a 4, indicativi di una situazione sanitaria compatibile con l'assolvimento del servizio militare quale volontario in ferma prefissata di un anno con limitazioni e con l'esclusione, in ogni caso, dall'impiego in operazioni fuori area e nelle zone a rischio malarico, tipologia che in ragione della natura dell'impiego dei militari con il nuovo sistema puramente professionale è evidentemente estremamente penalizzante. Quindi, da un lato è vero che la commissione scientifica nel suo documento conclusivo ha affermato che il deficit in questione «non può essere considerato fattore di discriminazione nella valutazione medico-legale dell'idoneità al servizio militare», dall'altro la stessa commissione ha però individuato le due predette classi di soggetti fabici, definendone i valori di riferimento e ritenendo idonei al servizio militare incondizionato i soli soggetti appartenenti alla prima classe ed idonei al mero servizio militare (dunque non incondizionato) quelli appartenenti alla seconda. La Difesa, comunque, per nulla insensibile alla problematica, tiene la stessa nella massima considerazione, ben consapevole di quanto sia importante dare una risposta certa e definitiva a tutti quei giovani che aspirano ad arruolarsi nelle Forze armate. Proprio nell'ottica di armonizzare i criteri di idoneità con i prevedibili progressi e scoperte nel campo medico-scientifico, la materia continua ad essere oggetto di particolare attenzione da parte degli organi sanitari del Dicastero che hanno, tra l'altro, già avviato contatti con l'Organizzazione mondiale per la sanità al fine di appurare se esistano varianti dei ceppi di malaria che sembrerebbero essere presenti in alcune aree di prevalente impiego operativo per il personale delle Forze armate. Devo far presente, tuttavia, che nei bandi di reclutamento di volontari di truppa in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate, banditi dalla competente Direzione generale per il personale militare, è prevista, anche per il 2010, l'esclusione dall'ulteriore *iter* concorsuale dei candidati che, al termine degli accertamenti sanitari, siano stati riconosciuti affetti da patologie, in generale, per le quali è prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, indipendentemente quindi dalla tipologia di imperfezione o di infermità. Ciò, fermo restando l'autonomia di ogni Forza armata, in quanto il quadro giuridico vigente attribuisce direttamente ai Capi di Stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la competenza ad ad emanare direttive per il reclutamento e la selezione del personale, attraverso l'individuazione di specifici requisiti psicofisici relativi alle diverse esigenze di impiego. Con particolare riferimento, invece, ai soggetti fabici, vorrei ulteriormente chiarire che l'esclusione dalle procedure concorsuali dei candidati affetti da deficit G6PD con coefficiente del profilo sanitario pari a 3-4 non è riconducibile semplicemente alla carenza di tale enzima in senso assoluto, ma è prevista unicamente, allo stato attuale, per quei soggetti la cui carenza risulta essere superiore ai livelli percentuali individuati dalla commissione scientifica, fermo restando l'inidoneità al servizio militare per i soggetti con «deficit di G6PD che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche». Tale limitazione è finalizzata a garantire la salute dei soggetti affetti da favismo che, pur con tutte le precauzioni d'impiego, potrebbero essere esposti, per cause imponderabili, al rischio di crisi emolitiche gravi. Infatti, premesso che la carenza di G6PD, in assenza di fattori esterni che determinano un danno ossidativo a carico dei globuli rossi, non corrisponde ad uno stato di inabilità, pur tuttavia, ove esistono una predisposizione e il rischio di crisi emolitiche anche episodiche, è indispensabile garantire l'applicazione di adeguate misure preventive. In ultimo, rammento che sono in corso di esame alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare:

*(PdL)*. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Cossiga per la sua risposta. L'esclusione dei soggetti fabici dall'arruolamento nelle Forze armate è una questione che interessa moltissimo i giovani che vorrebbero intraprendere la carriera militare. Il deficit enzimatico relativo al cosiddetto G6PD riguarda infatti circa 400.000 italiani, ma, mentre nelle altre Regioni interessa un'esigua parte della popolazione (dall'1 al 7 per cento dei giovani sardi (la mia terra, la sua terra, signor Sottosegretario) ne è affetto. Conseguentemente, molti ragazzi della nostra Regione si vedono ingiustamente esclusi dalla possibilità di arruolarsi nelle Forze armate. Nonostante la carenza enzimatica sia abbastanza diffusa, gli episodi di crisi emolitiche acute sono molto limitati. La stragrande maggioranza dei fabici non sa nemmeno di esserlo: conduce una vita normale ed è abile ad eseguire qualunque lavoro. Dopo l'emissione delle risultanze della commissione scientifica e la modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di fatto sussistono ancora alcuni fattori ostativi che impediscono a molti giovani fabici di indossare la divisa. Dopo le tante battaglie politiche e giudiziarie potremmo finalmente scrivere le parola fine su questo problema solo rimuovendo questa antica discriminazione a danno di tantissimi giovani. Mi dichiaro

mi riferisco all'interrogazione della senatrice Blazina e di altri senatori con la quale si chiedono informazioni circa gli interventi del Ministero in favore del Teatro stabile in lingua slovena. A tale proposito, voglio anzitutto rappresentare che il Ministero per i beni e le attività culturali è a conoscenza della situazione di crisi del teatro, situazione che, però, va ricondotta esclusivamente ai rapporti tra lo Stabile e le autonomie locali e in relazione alla quale vi è, comunque, già stato un intervento statale a livello locale che ha coinciso con l'attività di coordinamento svolta dal prefetto di Trieste nei confronti dei soci enti locali. Per quanto riguarda gli interventi diretti del Ministero, voglio in particolare evidenziare che il supporto finanziario allo Stabile in lingua slovena è sempre stato costante e che, nell'anno 2009, nonostante la diminuzione di circa il 6 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo per gli stabili pubblici, il contributo al teatro in argomento ha subito una decurtazione di solo il 3 Ciò premesso, ritengo opportuno far presente che la nuova stagione 2009-2010 è comunque partita e che, pertanto, i timori di interruzione dell'attività espressi nell'interrogazione non hanno avuto riscontro. Infine, in merito a quanto espresso dalla senatrice interrogante circa la necessità di ricercare soluzioni strutturali nell'ambito delle norme e dei regolamenti applicativi sui teatri stabili, devo rappresentare che le relative disposizioni statali incidono in misura assai limitata sulla tipologia di struttura di struttura giuridica adottata dal teatro nonché sui contratti privati che vengono stipulati fra gli stabili pubblici e tutte le varie figure professionali coinvolte nella produzione artistica. Pertanto, ritengo che non esista ulteriore spazio per un intervento statale, atteso che gli stabili pubblici godono già dell'autonomia necessaria per individuare le forme contrattuali più efficienti.

di Slovenia e ulteriori finanziamenti degli enti locali, che fino a quest'anno non erano conseguenti agli impegni assunti, essendo gli enti locali soci fondatori del Teatro.

per la sorte del Teatro nei prossimi anni in relazione a queste difficoltà strutturali. Nella mia interrogazione volevo far presente al Ministero competente che ulteriori riduzioni del FUS andrebbero certamente a peggiorare la situazione del Teatro sloveno, e quindi vi è

si possa trovare una soluzione, nella convinzione che questo Teatro, oltre ad essere l'ente culturale di eccellenza per la comunità slovena, è anche un ente culturale

mi riferisco all'interrogazione del senatore Latronico riguardante la proposta di vincolo paesaggistico del territorio comunale di Irsina ai fini dell'adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico. In merito voglio portare a conoscenza del senatore interrogante le varie fasi e lo stato attuale del procedimento, svolto finora dai diversi uffici del Ministero competenti per materia. In data 17 ottobre 2008 la Soprintendenza, al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse paesaggistico del territorio in questione, in considerazione della rilevanza dei valori paesaggistici e culturali da esso espressi, ha proposto alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata l'adozione del provvedimento di vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 138 del codice dei beni culturali. Successivamente, in data 30 luglio 2009, la predetta proposta è stata inoltrata alla Regione Basilicata per acquisire eventuali preliminari osservazioni in merito. Trascorso infruttuosamente il termine di trenta giorni prescritto dall'articolo 138, comma 3, del codice, la predetta direzione regionale ha ritenuto di dover procedere in via surrogatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 141 del citato codice, avviato il procedimento trasmettendo, in data 14 settembre 2009, la proposta di vincolo al Comune di Irsina per la sua pubblicazione e provvedendo, contestualmente, a darne notizia sui siti informatici e sui quotidiani a tiratura regionale e nazionale per le previste osservazioni degli enti territoriali e degli aventi causa. A seguito di una preliminare istruttoria, la citata direzione regionale, su richiesta della Direzione generale per il paesaggio, ha inviato, in data 4 dicembre 2009, una documentazione integrativa al fine di precisare le prescrizioni di tutela dettate nella proposta di vincolo. Ciò premesso, voglio rappresentare che, allo stato attuale, la competente Direzione generale ha precisato alla predetta direzione regionale come siano opportune l'elaborazione della documentazione e l'individuazione grafica dei beni e dei perimetri delle aree indicate. Per quanto riguarda, infine, le considerazioni formulate dal senatore interrogante sull'opportunità o meno di adottare il provvedimento di vincolo paesaggistico nonché sulla ridefinizione delle aree da sottoporre ad esso, voglio far presente che gli uffici territoriali del Ministero, nel ribadire come il territorio in argomento appaia meritevole di tutela in considerazione delle sue molteplici peculiarità, hanno comunque assicurato la disponibilità a valutare le proposte di ridefinizione delle zone che verranno formulate dagli enti territoriali in sede di acquisizione delle osservazioni di cui al comma 5 dell'articolo 139 del codice. **Saluto

vi è stata una certa sollecitazione a valutare in maniera più dettagliata l'imposizione del vincolo paesaggistico sull'intero territorio comunale, anche su aree che, su aree che, a detta dell'autorità locale, non avrebbero le caratteristiche e il pregio che sono il presupposto della tutela paesaggistica. Questo, ovviamente, per le implicazioni che l'imposizione del vincolo paesaggistico poi poi comporta sulle attività presenti sul territorio: mi riferisco in modo particolare alla presenza di aree industriali e di aree con intensa attività agricola, che sarebbero state tutte incluse all'interno della prima proposta di vincolo. Quindi, il senso dell'interrogazione andava nella direzione che mi sembra di cogliere nella risposta del Sottosegretario. Aggiungerei solo

possa pervenire a definire quelle realtà territoriali che hanno necessità di tutela senza porre un vincolo indiscriminato, che finisce proprio

Con riferimento all'interrogazione dei senatori Lannutti e Giambrone con la quale essi chiedono informazioni sulla situazione riguardante lo sfratto dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, voglio rappresentare lo svolgimento dei fatti succedutisi nel tempo, che dimostrano tutti gli sforzi compiuti dal Ministero per i beni e le attività culturali al fine di arrivare ad una soluzione della vicenda. La situazione conflittuale dello sfratto dell'Istituto è venuta a precipitare nel mese di gennaio 2008 allorquando perviene al Ministero la richiesta di documentazione da parte dell'Avvocatura generale dello Stato affinché si possa procedere alla difesa in giudizio dell'amministrazione contro contro l'intimazione per finita locazione alla data del 31 dicembre 2008 e contestuale citazione per la convalida di sfratto. L'amministrazione ha immediatamente provveduto a comunicare alla proprietà di essere intenzionata a lasciare l'immobile, compatibilmente con i tempi necessari alla realizzazione dei lavori di restauro dei nuovi locali, individuati nell'ex carcere del Complesso del San Michele, che dovrebbero ospitare l'Istituto centrale del restauro. Pertanto è stata chiesta una ulteriore proroga della locazione alla controparte che, però, all'udienza del 28 gennaio 2008, manifestava l' indisponibilità ad un rinvio dello sfratto. Conseguentemente il giudice civile di Roma, con ordinanza del 12 febbraio 2008, ha convalidato la licenza di finita locazione al 31 dicembre 2008, fissando la data del 31 gennaio 2009 per l'esecuzione del rilascio. Nel frattempo, il Ministero ha informato l'Agenzia del demanio circa la convalida della licenza di finita locazione, facendo presente la volontà dell'amministrazione di insistere con la controparte per avere una proroga quinquennale della locazione per il periodo necessario alla realizzazione dei suddetti lavori di restauro ed adeguamento dei nuovi locali. Nel contempo, si chiedeva all'agenzia di porre in essere i provvedimenti di competenza ai fini della quantificazione del canone congruo e del prescritto rilascio del nulla osta alla spesa. In data 23 ottobre 2008, l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro ha nuovamente interessato l'Agenzia del demanio per ribadire la volontà di liberare l'immobile chiedendo di verificare la disponibilità di un edificio demaniale adeguato alle esigenze funzionali dell'Istituto, senza oneri di spesa per il Ministero. Tra i mesi di gennaio e febbraio 2009, a seguito della notifica dell'atto di intimazione per il rilascio dell'immobile nel termine di dieci giorni dalla data del 31 gennaio 2009 e di procedere ad esecuzione forzata, veniva intrapresa una intensa trattativa tra il Ministero e la Congregazione proprietaria, al fine di trovare un accordo con la controparte finalizzato alla predetta proroga per la durata di quattro-cinque anni ad un canone finanziariamente sostenibile e che tenesse conto delle ingenti spese sostenute dal Ministero negli anni per i lavori di consolidamento, restauro ed adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro effettuati sull'immobile. Il canone proposto, corrispondente al valore di mercato, era sensibilmente inferiore a quello richiesto dalla Curia generalizia e, pertanto, le trattative non sono andate a buon fine. Successivamente, in data 12 febbraio 2009, l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro ha esposto all'Agenzia del demanio, pur ritenendola giuridicamente insostenibile, la richiesta avanzata dalla Confraternita di poter acquisire Sant'Andrea delle Fratte in cambio di una proroga del contratto di locazione ad un canone aggiornato.

ha predisposto un contratto di locazione passiva volto a definire tutto il contenzioso pregresso e a disciplinare il rapporto locativo per la durata di quattro anni. La Congregazione ha però respinto la proposta arroccandosi su una posizione di totale chiusura ed impedendo una definizione conciliativa della vicenda. Di fronte a questo atteggiamento della Congregazione ed a seguito della nuova intimazione comunicata dall'ufficiale giudiziario per la esecuzione dello sfratto prevista per il 28 gennaio 2010, già dal mese di ottobre 2009 il Ministero si è attivato per dar corso all'unica soluzione possibile rimasta e, cioè, intensificare i lavori in corso nel Complesso del San Michele al fine di trovare una collocazione al personale ed agli uffici dell'Istituto sfrattati. Sulla base dei fatti riportati, ritengo di dover evidenziare che il Ministero ha messo in campo tutte le energie e soluzioni possibili per addivenire ad un accordo definitivo in tempi ragionevoli con la Congregazione che tenesse conto sia delle richieste dei Padri, sia delle ingenti somme sostenute dall'amministrazione negli anni per i lavori necessari di adeguamento e messa in sicurezza dell'immobile e sia delle risorse finanziarie a disposizione. Voglio comunque rappresentare che il Ministero per i beni e le attività culturali, per far fronte alle conseguenze della chiusura della Congregazione ad ogni margine di trattativa, è tuttora impegnato in un complesso lavoro di recupero e ristrutturazione degli spazi disponibili presso il Complesso del San Michele. A tal proposito, comunico che con decreto ministeriale 19 gennaio 2010 sono stati approvati, nell'ambito della programmazione triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i predetti lavori di restauro e adeguamento locali necessari per la sistemazione dell'Istituto. Infine, ho il piacere di comunicare che proprio nella giornata di ieri è stato sottoscritto un accordo tra l'amministrazione e tutte le organizzazioni sindacali interessate con il quale si prevede che l'Istituto superiore del restauro ritorni nei locali originariamente destinati all'istituto ai tempi di di Giovanni Urbani nel Complesso di San Michele, con accesso da piazza di Porta Portese. In tal modo, pertanto, il Ministero realizzerà importanti risparmi di spesa sui canoni di locazione prima corrisposti e nello stesso tempo l'Istituto disporrà di una sede prestigiosa, definitiva e idonea a soddisfare tutte le sue esigenze funzionali. La complessa e annosa questione, quindi, è stata chiusa e risolta.

accade che proprio il Ministero per i beni e le attività culturali, pur disponendo di beni considerevoli e di un patrimonio immobiliare

dal Ssttosegretario, onorevole Giro, nella risposta, che consideriamo soddisfacente. Ma questo la dice lunga sul rimpallo ricorrente delle responsabilità. L'Italia è un Paese che ha poco petrolio.

il cinquecentesco palazzo Borgia Cesarini e una parte del convento seicentesco annesso e a curarne l'allestimento e l'adeguamento funzionale per realizzare la sua pionieristica idea di istituto multidisciplinare. Nel corso degli anni cospicue risorse economiche dello Stato sono state impiegate per la conservazione e l'ammodernamento tecnologico di ambienti ed impianti indispensabili per la finalità di ricerca, formazione e restauro che l'Istituto da sempre svolge in Italia e nel mondo,